nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del disegno di legge, composto del solo articolo 1. È iscritto a parlare il senatore Allocca. Ne ha facoltà. Signor Presidente, ringrazio lei e anche i presenti, sebbene pochi, che oggi ci permettono di non essere in perfetta solitudine. Si parla con difficoltà per i posteri; è meglio invece interloquire tra noi e forse è anche più produttivo. più produttivo. Infatti il conflitto è il sale della democrazia: dentro e fuori quest'Aula attraverso il confronto e anche lo scontro - naturalmente mi riferisco a quello dialettico - noi stessi, e con noi i cittadini che abbiamo il dovere e l'ambizione di rappresentare, compiamo quel necessario percorso di comprensione della realtà e di sistemazione organica e coerente dei fatti che ci consente di operare scelte consapevoli, non affidandoci di volta in volta all'umore mattutino. Oggi a me sembra che sia in scena qualcosa che in apparenza scombina questa sistemazione organica. Io che sono un comunista non pentito, oggi mi trovo a difendere un provvedimento con un impianto sostanzialmente liberale; dall'altra parte, invece, una compagine che si autodefinisce Casa delle Libertà, riferendosi essenzialmente a quelle economiche, lo osteggia fortemente. circostanza merita qualche considerazione generale - seppur breve nei pochi minuti che ho a disposizione - che non può essere elusa e non riguarda nemmeno gli equilibri interni della coalizione di Governo, né le categorie, pure nobili, della mediazione e dell'affidabilità politica, ma riguarda, a mio avviso, una degenerazione che ha investito la stessa economia di mercato a cui è comunque necessario mettere mano dall'interno di quelle logiche. Viviamo un tempo, signor Presidente, in cui l'offerta non è più in equilibrio con la domanda, come recitano i classici, ma la governa in modo assoluto; un tempo in cui i bisogni primari e anche il malessere sociale vengono occultati, digeriti e trasformati in desideri immediati di merce, dove la pubblicità e le promozioni commerciali non ti dicono più cosa devi comprare, ma come devi essere: *homo acquirens*, magari povero, ma sempre e comunque consumatore. Per questa via, quello che i lavoratori percepiscono (poco in verità, come ci dicono anche le statistiche recentemente pubblicate, che collocano l'Italia al penultimo posto per quanto riguarda il potere d'acquisto di salari e pensioni), questo scarso salario viene rapidamente drenato e torna alla casa madre del grande capitale proprio attraverso l'incentivazione al consumo. Penso ai ragazzi delle scuole medie, che incontro la mattina in autobus quando vengo in Senato, figli di lavoratori che alle 8 della mattina già fumano e fanno colazione con i telefonini in mano. I telefonini, la nuova merce virtuale, il surrogato informatico della piazza dimenticata dall'urbanistica moderna, una comunicazione ossessiva e compulsiva come contraltare di una dilagante solitudine esistenziale. Per questo l'articolo 1 del decreto che oggi viene convertito in legge a me sembra un qualcosa di sinistra e non solamente perché, indipendentemente dalla sua entità economica, si pone comunque

promuovere una diversa modalità dell'offerta, caratterizzata da una maggiore trasparenza e da una minore induzione al consumo. Non a caso, su questo articolo si è molto dibattuto in Aula e in Commissione, con diverse argomentazioni. È stato detto che con tutta probabilità le compagnie telefoniche recupereranno la perdita subita per l'eliminazione dei costi fissi di ricarica sul traffico reale, riversandola sul costo della chiamata. Può essere che sia così, anche se non avverrà immediatamente; ma intanto viene cancellata una pesante ingiustizia, che faceva pagare di più a chi aveva meno da spendere, che gravava consistentemente sulla scheda da dieci euro (quella che acquistano studenti e immigrati), una diversa relazione tra domanda ed offerta che non abbia al centro esclusivamente la spinta al consumo. Su questo come sugli altri singoli provvedimenti relativi alle assicurazioni, ai mutui, alle compagnie *low cost*, si poteva forse fare meglio. Certamente a questo avrebbe anche contribuito un confronto aperto e di merito, signor Presidente, che non si è potuto realizzare, in parte per una responsabilità, dal nostro punto di vista oggettiva, realizzata alla Camera e in parte, invece, per un'impossibilità che si è determinata in quest'Aula. colleghi, questo confronto, che, come dicevo, non si è voluto fare alla Camera e non si è potuto fare al Senato, ha determinato un'incapacità di un approfondimento e ci sono state critiche, comunque rinnovate anche qui in quest'Aula, nei confronti della minestra che il centro-sinistra ha cucinato, con osservazioni, per la verità, molte volte contrastanti: era troppo salata, era poco salata; fuori di metafora, era troppo statalista o troppo liberista; era troppo poca o troppa. Non è un caso, però, che quando noi siamo arrivati, signor Presidente, la cucina era fredda e il fuoco era spento. Ho l'impressione che il problema sia proprio - e questo richiama quel dubbio da cui eravamo partiti - che questa minestra e questo approccio forse mancano totalmente nel menu e nelle prospettive della Casa delle Libertà, quindi chiudiamo la nostra argomentazione confortandoci su tale questione. Devo intervenire a difesa della minestra, colleghi, perché è sempre utilizzata in termini di confronto negativo, quando invece ci sono delle ottime minestre! È iscritto a parlare il senatore Baldassarri. Ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo provvedimento si completa il quadro della politica economica dell'attuale Esecutivo nel suo primo tormentato anno di governo. Se ripercorriamo gli elementi essenziali e portanti della strategia di politica economica, e se dovessimo giudicarla sulla base delle regole con le quali si giudicano i bilanci di impresa e le relazioni delle imprese, cioè sulla base del buon senso, dovremmo concludere che questa strategia e questo primo tormentato anno di governo, nel quale si è già succeduto un Governo Prodi-*bis* fotocopia, si caratterizzano per tre reati: false comunicazioni sociali, falso in bilancio e abuso di titolo dei decreti e delle leggi. Ovviamente, in quest'Aula non troppo piena, nella sordità dei *mass* *media,* tre reati possono anche essere considerati delle assurdità di un individuo che li segnala. C'è un aspetto istituzionale profondo nella politica economica del Governo, centrata su tre reati: false comunicazioni sociali, falso in bilancio e uso abusivo di titoli nei decreti e nelle leggi. Ma, a ben vedere, l'origine di tutto questo è il cancro genetico che alla nascita ha caratterizzato questa maggioranza e questo Governo. Non essendo d'accordo su nulla, qual è la conseguenza nell'operare concreto dell'azione di governo? conseguenza è che all'interno di questa maggioranza gli accordi si possono trovare sulla base di manifesti ideologici, come ad esempio per i DICO, che non a caso scontentano l'una e l'altra parte; puri manifesti ideologici, perché in tema di diritti soggettivi

dei conti: lo ripeto ancora una volta, alla luce della trimestrale di cassa, presentata dal Ministro dell'economia, dal quale ancora la Commissione e l'Assemblea attendono risposte rispetto alla contabilità del bilancio dello Stato, e alla luce di qualche vaga interpretazione di pseudoesperti che si firmano sulla stampa quotidiana con il nome delle istituzioni (uno SECIT, un altro Ministero dell'economia e delle finanze, e c'è da chiedersi se questi signori, scrivendo sui giornali, hanno titolo per parlare sul piano personale o sul piano istituzionale) il bilancio dello Stato di quest'anno il bilancio dello Stato di quest'anno è falso. Non solo mancavano 23 miliardi delle entrate 2007 sulla base dei risultati consuntivi delle entrate 2006 (23 miliardi era la contabilizzazione quando a dicembre il Governo si basava correttamente su ipotesi di crescita economica minori di quelle che si sono rivelate) ma a marzo, nella trimestrale, nel momento in cui il Governo indica una crescita del 2 per cento nel 2006 e del 2 per cento nel 2007, il falso in bilancio si quantifica in 26 miliardi di euro.

per non toccare gli anelli grossi e pesanti che stanno a monte di quella filiera di incrostazioni di poteri oligopolistici e, per agevolare anzi, come risultato finale, il rafforzamento di quei poteri, possibilmente amici. Vado solo per titoli. Per i tassisti, il provvedimento originario prevedeva addirittura la possibilità che alcune grandi imprese multinazionali o grandi cooperative potessero accedere, a colpi di 500-1.000 licenze con l'intento di sostituire a lavoratori autonomi, i cosiddetti padroncini, delle grandi organizzazioni multinazionali o delle grandi cooperative, trasformando i lavoratori autonomi in lavoratori dipendenti, magari

quota fissa sul telefonino. Collega Allocca, non lo dicono le previsioni, lo ha detto formalmente il Governo che si determinerà - parole del Governo in Commissione - una ristrutturazione delle tariffe e un aumento del traffico, per cui non diminuirà il fatturato delle aziende e, di conseguenza, non diminuirà il gettito. Il Governo ha fatto un autogol clamoroso: nel tentare di rispondere al dubbio circa la presenza di un problema di copertura di gettito a seguito della cancellazione della quota

tutto ciò non è affatto casuale: c'è dietro un preciso disegno strategico, ognuno per il proprio ruolo e la propria C'è chi vuole favorire le concentrazioni bancarie, chi le concentrazioni delle cooperative e magari c'è chi vuole favorire alcuni grandi gruppi multinazionali che dominano la grande distribuzione del Paese. Quello che mi meraviglia, collega Allocca, è il fatto che proprio la sinistra cosiddetta alternativa, succube di questo disegno strategico, o non vede o fa finta di non vedere di essere strumento non per le liberalizzazioni,

della costituzione di grandi concentrazioni di potere che tali sono, anche quando si chiamano cooperative rosse. *(Applausi

Il 25 luglio si è svolta in quest'Aula un'ulteriore discussione su un primo pacchetto di provvedimenti; ricordo che allora i giornali e alcuni esponenti del centro-destra avanzarono considerazioni del tipo: abbiamo dovuto aspettare altri per fare quel che avevamo detto di voler fare noi. Stiamo parlando di misure serie, che giovano al Paese e che, se attivate nel modo migliore possibile, ci riagganciano a dei filoni che avevamo perso in passato, ad onta della dichiarata e manifestata volontà liberale della precedente maggioranza. un tema sul quale è del tutto evidente che discussioni come quella di tipo domestico di questa mattina a ben poco servono. Noi dell'Italia dei Valori daremo il voto di fiducia al Governo, però non possiamo non rimarcare le modalità con cui si procede su una questione così importante, come ho già sottolineato. È del tutto sbagliato non ragionare compiutamente su una di quelle che saranno le strutture portanti della nostra economia. È del tutto sbagliato concentrare in pochissimi minuti l'attenzione su provvedimenti che segnano profondamente - e dal nostro punto di vista profondamente in positivo - la vita dei cittadini. Liberalizzare, lungi dal pensare

mettendo al centro il cittadino e non più gli interessi di altri, quindi gli interessi del cittadino e tutto ciò che si muove intorno visto in funzione degli interessi del cittadino stesso. E non è poco. Se non è poco, allora stiamo probabilmente sbagliando a discutere in questo modo, perlomeno qui al Senato.

Se qualcuno ha deciso che stiamo diventando una democrazia monocamerale, ha il dovere di dirlo nelle sedi competenti, in modo da poter realizzare le riforme costituzionali che portano a ciò. Fin quando così non sarà, ogni Camera ha il dovere, perché siamo pagati dai cittadini per fare ciò, di esaminare compiutamente i provvedimenti da adottare, soprattutto quando tali provvedimenti vanno a incidere sulla sfera dei diritti del cittadino, ossia dei nostri datori di lavoro. datori di lavoro. Il presidente Marini lo ha detto, ma credo che la Presidenza e tutte le forze politiche si debbano far carico dell'esigenza di un'armonizzazione vera rispetto alla possibilità di esame dei provvedimenti da parte delle due Camere. Siamo ancora in un sistema di bicameralismo perfetto ed è bene che ogni parlamentare possa esercitare le sue prerogative. Faccio solo un esempio di quanto avrei voluto dire se ce ne fosse stata la possibilità. Parliamo Parliamo delle assicurazioni. Oggi molti di noi hanno un'assicurazione sulla vita non disdettabile. Che cosa succede se uno di noi che ha un'assicurazione sulla vita non disdettabile è colpita da un infarto? infarto? Che l'anno successivo, probabilmente, l'istituto assicurativo disdetterà, perché si libera dal rischio di aspettare fin quando non va a scadenza la polizza. Abbiamo riflettuto su questo fatto? Possiamo rifletterci in pochi minuti?

Oggi il Governo otterrà la fiducia da questa Camera, ma la Presidenza del Senato ha il dovere di porre con forza e fermezza - e tutte le forze politiche hanno il dovere di sostenere questo tentativo - il fatto che tutti i parlamentari, e quindi anche i senatori, hanno il diritto di esaminare compiutamente i provvedimenti che devono votare.

Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, unitamente alle questioni sulle quali si è già soffermato il senatore Formisano e che condivido, devo dire che questa fiducia è la prima che mi sento di dare con convinzione. Esistono questioni che possono essere utilizzate in chiave non completamente positiva. Del resto, pur sentendomi un riformista, provengo dall'esperienza comunista e di sinistra dove il termine liberalizzazioni nell'esperienza maturata - visto che di anni ne ho messi assieme mi dice che liberalizzare è dare libertà al forte, togliere libertà al debole, oppure libera volpe in libero pollaio. Quindi, quando si parla di liberalizzazioni mi

a tutta la sinistra, ma anche al Gruppo Misto, al quale mi onorerò di porre la questione, di sviluppare ulteriormente il tema della partecipazione dei consumatori.

di elementi positivi ma - come dire - non abbiamo ancora morso la polpa per quanto riguarda le banche. Siamo tutti in Europa, tutti abbiamo l'euro, ma in Italia il costo del denaro va dall'1,5 al 2,5 in più per i consumatori. Quindi, il grande tema della presenza dei consumatori deve essere affrontato. Propongo al Governo di lavorare per dare vita ad un vero e proprio statuto dei diritti dei consumatori perché nessuno si senta solo di fronte all'arroganza e alle ingiustizie degli strumenti pubblici

colleghi senatori, in premessa intendo confermare la nostra opinione positiva sul decreto Bersani, oggi chiamati a difendere con il voto di fiducia. Questa nuova ondata di liberalizzazioni, sintetizzando le varie segnalazioni dei privati e delle associazioni, si è concentrata sul cittadino consumatore al fine di liberare energie e risorse di crescita del Paese. Perciò, va apprezzata come manovra volta ad incentivare lo sviluppo economico del Paese, abbattendo barriere poste da un'economia protezionistica. È un momento delicato in cui non si può gridare al «finto liberismo»

liberalismo è ideologia politica democratica. Entrambi, per essere al passo con i tempi, devono coincidere per fondare l'essenza di uno Stato in cui democrazia voglia dire libertà economica. Le due regole, che sostengono il disimpegno dello Stato ed esaltano l'individualità nel mercato, devono spontaneamente evolvere verso la struttura economica più efficiente possibile, che sia il «mondo migliore per produttore e consumatore». Né l'una, né l'altra può appartenere a chi si compiace nel definirsi liberista, ma fa battaglie e obiezioni scatenate contro questo decreto-legge: costui non aiuta l'Italia a crescere. Perciò sanno di ipocrisia le doglianze di parzialità rivolte alla manovra, né sono legittime le insulse critiche di carenza di gradualità, perché vanno contro gli interessi del Paese. Con il decreto-legge Bersani, infatti, il Governo, ha dato un deciso segnale di apertura del mercato ed ha realizzato la spinta europeista che ci insegna a garantire la libera concorrenza e ad annullare gli ostacoli allo sviluppo economico. La manovra delle liberalizzazioni, quindi, realizza il *diktat* comunitario e si riflette su molteplici settori strategici per i cittadini-consumatori abbattendo vincoli amministrativi, improntando il mercato verso un ordine crescente che associ la nozione di libero scambio ad un'economia globale lontana da un'obsoleta visione protezionista. In tal senso si leggono le disposizioni relative all'abolizione dei costi fissi di ricarica dei cellulari, alle autocertificazioni, alle norme del plurimandato assicurativo, come tutte quelle concernenti le agevolazioni dei mutui. I provvedimenti contenuti nel decreto-legge in esame, secondo le associazioni dei consumatori, incidono, peraltro, per un giro d'affari di oltre 22 miliardi di euro e, quindi, oltre a migliorare la qualità dei servizi in un mercato più trasparente, possono realizzare oltre 1.000 euro l'anno di risparmio per ogni famiglia. Dunque, non si può sottovalutare l'incidenza positiva delle modifiche normative che disciplinano vari settori il cui sviluppo accresce il sistema produttivo nazionale ed incentiva il progresso economico. Di qui l'urgenza di approvare il provvedimento in esame, che palesa il nesso di funzionalità con l'indirizzo politico del Governo di modernizzazione del sistema produttivo e di snellimento delle procedure burocratiche. Pertanto, quest'oggi i Popolari-Udeur confermano la fiducia al Governo Prodi sul provvedimento in oggetto.

i molti motivi di critica e di perplessità legati, oltre che al contenuto, al metodo che è stato adottato per invitarci a dare il nostro contributo nella formazione di questa legge. Ebbene, abbiamo criticato tutti l'uso reiterato del voto di fiducia, ma soprattutto il metodo della decretazione d'urgenza per risolvere problemi che avrebbero potuto trovare ampio spazio e più comoda trattazione in quest'Aula. Certamente, stiamo scivolando verso una china pericolosa

del voto di fiducia finisce per togliere validità al lavoro di entrambe le Camere. Si tratta, quindi, di un metodo antidemocratico. Sono molto soddisfatto che anche dall'altra parte dell'emiciclo si levi qualche voce di critica a questo metodo. Del resto, devo riconoscere con onestà che ieri il ministro Chiti, nell'annunciare l'apposizione della fiducia, non ha nascosto un certo imbarazzo che, nel mio infinito buonismo, voglio anche immaginare sincero, attribuendo questa soluzione al prolungamento del dibattito alla Camera dei deputati e, quindi, alla necessità di pervenire all'approvazione del provvedimento al Senato entro i termini di scadenza, ormai imminente. Il ministro Bersani, invece, è stato molto più esplicito e forse anche ingeneroso parlando direttamente di ostruzionismo praticato dai deputati della Casa delle libertà, e annunciando con toni molto calorosi

una graziosa concessione della maggioranza e non un diritto, una prerogativa irrinunciabile di tutti parlamentari. Inoltre, il ministro Bersani - è un peccato parlare sempre in assenza degli interessati - con il suo tono di ben noto affabulatore ci ha invitati al dialogo

- mi sia consentita un'amara allegoria - a parlare e a dialogare con un bavaglio sulla bocca, a scrivere emendamenti con le mani legate dietro la schiena

perché in fondo questa legge, accanto a molti aspetti criticabili, contiene anche qualche proposta condivisibile. La parte condivisibile riguarda sicuramente gli interventi di minore spessore, che coinvolgono categorie alle quali va - per carità - tutto il nostro rispetto: le guide turistiche, i barbieri, i parrucchieri, i panificatori, le autoscuole, gli addetti alle attività di facchinaggio, gli acconciatori, le estetiste, gli operatori nel settore della pulizia e della disinfezione. Le soluzioni

il problema del nostro prodotto interno lordo sia nei rapporti con l'Europa che a livello interno. E poi, tutte queste liberalizzazioni, in fondo, appartengono alla pratica quotidiana dei rapporti con le camere di commercio, oppure alle competenze dei Comuni e delle Province. Per quanto riguarda gli altri aspetti maggiormente di sostanza, molti si sono soffermati, giustamente, su settori più importanti, come quello delle grandi opere, la TAV, la telefonia, i servizi Internet, il mercato delle comunicazioni in generale, come pure sul sistema di rifornimento di carburante in autostrada e così via. Anche sul mercato del gas c'è una citazione ed è un po' strano, in quanto

In molti casi, inoltre, si interviene a gamba tesa sulle regole del libero mercato e molte norme potrebbero essere impugnate in quanto incompatibili con i principi del mercato unico europeo. Gli esempi sono stati fatti durante la discussione generale. Tutti hanno citato il settore della telefonia mobile. Siamo tutti d'accordo sulla sulla soppressione dei costi fissi, sui costi di ricarica e su tutto quanto va a favore del consumatore, ma molti colleghi esperti hanno già indicato gli *escamotage* che saranno messi in atto dalle società per recuperare questo eventuale divario. Va detto che il popolo di Internet si è già attivato. Ho qui una *e-mail* - l'avrete ricevuta in cui si annuncia una possibile ritorsione attraverso l'introduzione di una segreteria telefonica non richiesta, ma vi sono indicazioni su come disinnescare questa "bomba" prima che venga fatta esplodere. Vorrei ricordare che oggi sui giornali, sul tema della telefonia, c'è un richiamo forte della commissaria europea Viviane Reding, che invita l'Italia ad una maggiore trasparenza nelle sue operazioni, soprattutto per quanto riguarda il sistema dei ricorsi. Per quanto concerne il prezzo dei carburanti, introdotta è un palliativo. In molti Paesi europei già esiste l'indicazione dei prezzi fuori delle stazioni di servizio e non credo sia una grande riforma. Ben venga, invece, una maggiore trasparenza nell'esposizione dei costi complessivi dei voli *low cost*; ma, signori del Governo, perché non intervenire anche su un altro aspetto del nostro rapporto con le compagnie aeree, limitando i costi eccessivi delle compagnie di bandiera, che continuano ad applicare prezzi di monopolio come se non vi fosse stata, almeno per loro, la liberalizzazione del settore del trasporto aereo? Nel comparto dei servizi assicurativi, ben venga dal mio punto di vista - so di essere in contrasto con alcuni miei colleghi e mi dispiace, ma non cambio idea - una maggiore considerazione del ruolo dell'agente assicurativo, vero operatore del mercato del mercato tra le compagnie e l'assicurato, vero garante di ciò che l'assicurato vuole sentirsi dire nei momenti di difficoltà, quando fisicamente non c'è la compagnia, ma è l'agente che risponde dei contratti. Complimenti per l'idea di aiutare il consumatore a rescindere quei contratti decennali che rappresentavano spesso delle gogne, in in fondo nemmeno ben conosciute. Molta gente firma un contratto e non si rende conto di vincolarsi per oltre dieci anni. Peccato che non abbiate avuto il coraggio di eliminare

Quanto alla prima, non si interviene con un emendamento su una riforma sofferta, discussa e approvata nella precedente legislatura. Sulla TAV, non è vero - come qualcuno ha affermato ieri che non esistono pericoli di esclusione dai finanziamenti europei. I gravi provvedimenti adottati, con la scissione dei contratti delle concessioni per le tratte Milano-Verona-Padova e Milano-Genova, sono solo esempi, palliativi. I veri problemi sono le reti collegate alle TEN, il grande reticolato di collegamenti ferroviari che l'Europa ha disegnato nel 1993 e che ha portato avanti finora con l'Italia, che si è impegnata al

domanda, i problemi che pesano sull'economia italiana sono gravissimi, sintetizzabili in due grandi questioni: la bassa competitività delle imprese nel raffronto europeo e il crescente debito pubblico. problemi frenano lo sviluppo della nostra economia. Basti pensare che il debito dello Stato è cresciuto a quasi 1.600 miliardi di euro, per i quali tutti quanti, a danno della comunità, spendiamo all'anno oltre 65 miliardi di euro di soli interessi passivi. Questi soldi potrebbero essere investiti per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Con la finanziaria, tanto criticata, questo Governo è riuscito ad affrontare il problema della continua espansione del *deficit* che ancora nel 2006 ha sforato il tetto del 3 per cento, raggiungendo una quota oltre il 4 per Fortunatamente, allo stato, la situazione dei conti pubblici italiani sta gradualmente migliorando: nel 2007, infatti, il *deficit* potrà essere contenuto entri i limiti previsti dall'Europa, tanto sotto il 3 la fase di emergenza é stata superata e, come ha stimato il ministro del tesoro Padoa-Schioppa nella sua ultima audizione al Senato, è ipotizzabile addirittura una crescita del prodotto interno lordo superiore al 2 Il problema del debito, però, deve rimanere sotto controllo per liberare risorse e favorire tutta la comunità. Per quanto riguarda invece il secondo problema di cui soffre l'Italia, cioè la mancata competitività delle imprese, servono ulteriori ed importanti riforme soprattutto aprendo e liberalizzando il mercato. Questa è la condizione propedeutica all'aumento della competitività: soltanto liberalizzando il mercato si favorisce l'iniziativa privata, si stimola il commercio e la concorrenza, anche perché la liberalizzazione è espressione evocativa dei bassi costi e dell'alta qualità e tutto ciò va a vantaggio dei cittadini in quanto consumatori. Questo Governo, già pochi mesi dopo il suo insediamento, ha dato con il primo decreto Bersani, in materia di liberalizzazione, un primo importante segnale perché ha messo mano dove finora nessuno ha osato. Con questo Con questo secondo decreto Bersani ritengo si aggiungano nuovi ed importanti passi al lungo cammino per la modernizzazione del nostro Paese. Le reazioni giustamente preoccupate delle categorie direttamente interessate dalle norme di liberalizzazione sono comprensibili, ma non devono scoraggiarci; infatti, non è più tollerabile che oggi, all'interno di un'economia sempre più aperta e globalizzata, l'Italia sia ancora dominata da un sistema corporativo che noi tutti rileviamo come del tutto anacronistico. Mi auguro intanto che gli oppositori abbandonino la loro attuale postazione di difesa di questi interessi corporativi che bloccano la crescita del nostro Paese. Loro stessi, invece, dovrebbero accettare le sfide che comunque il mercato globale ci pone davanti e contribuire a promuovere questo processo di modernizzazione e liberalizzazione. Solo anticipando i tempi di maturazione di questo processo e non subendo passivamente questo irreversibile processo, potranno attrezzarsi al meglio per fronteggiare una sempre più spietata concorrenza mondiale. Riteniamo che le misure contenute in questo decreto e nel disegno di legge che seguirà diano risposte concrete a questo bisogno. Tutto questo riguarda le imprese, ma liberalizzare significa anche creare più concorrenza, una maggiore e più qualificata offerta, più competitività e prezzi più accessibili, e tutto ciò va a vantaggio dei consumatori. Abbiamo già potuto constatare - i colleghi lo hanno già fatto i vantaggi di questo decreto per i consumatori: il divieto per le banche di far pagare la penale per l'estinzione dei mutui, la più semplice portabilità dei mutui da un istituto ad un altro, l'abolizione dei costi fissi per le ricariche dei telefonini (soprattutto i giovani ne saranno grati), costi fissi per le carte prepagate, per Internet e i programmi tv. Ricordiamo, inoltre, la modifica dei criteri d'attribuzione delle classi di merito per le assicurazioni RC Auto la maggior trasparenza nel settore assicurativo. Prima, anche il mio collega Santini ricordava la maggiore visibilità della data di scadenza dei prodotti alimentari e via dicendo. Sul fronte delle imprese c'è una grande semplificazione: d'ora in poi un'unica comunicazione sostituisce una serie di adempimenti burocratici per l'avvio di un'impresa. Questo è un grande passo avanti. Lo snellimento delle procedure è un indubbio vantaggio e uno stimolo per favorire nuove iniziative soprattutto da parte dei giovani che vogliono intraprendere un'attività. Oltre a ciò sono state eliminate per molti esercizi commerciali le limitazioni di orario ed i vincoli dettati dalle distanze minime tra negozi dello stesso tipo. Le imprese italiane, ne sono profondamente convinto, hanno bisogno di queste liberalizzazioni per aprirsi al mercato ed essere maggiormente concorrenziali e competitivi. É una sfida importante ma soprattutto necessaria per far sì che le nostre imprese riescano a tenere il passo delle imprese europee e mondiali, una sfida in un mercato globale che, se affrontata nella giusta maniera, darà all'intero Paese nuovo slancio e maggior benessere per tutti. Certo, e adesso vengo al secondo problema, il passaggio è molto delicato. Come dicevo all'inizio, si pone pertanto un'ulteriore domanda, come affrontare e governare le difficoltà che nascono da questo passaggio. Difatti, si passa da un sistema protetto e di mercato limitato ad una completa apertura, e non c'è dubbio che le nostre imprese sono nate e cresciute in un sistema basato su licenze, su concessioni, su protezioni: il sistema che nel passato limitava il loro raggio d'azione, li proteggeva da nuove concorrenze e li tutelava in ambito locale. Con le liberalizzazioni le stesse imprese si trovano davanti a uno scenario ed a coordinate completamente cambiati; pensiamo, ad esempio, ad un piccolo negozio, ad una farmacia, ad un benzinaio, ad una pensione o ad un artigiano di un piccolo centro. Secondo il sistema tradizionale questi dovevano investire, a suo tempo, ingenti somme non solo per l'avvio dell'attività ma spesso anche per l'acquisto di una licenza o di una concessione. Potevano però contare anche sul fatto che il piano commerciale, le licenze e così via gli garantivano una certa clientela. Domani lo stesso piccolo imprenditore si troverà di fronte ad un mercato aperto ed esposto alla forte concorrenza delle multinazionali. Servono pertanto, e questa è la mia conclusione, misure che promuovano le piccole e medie imprese per metterle in grado di affrontare queste sfide; bisogna aiutarle a crescere, ad aggregarsi, a sfruttare sinergie comuni, a specializzarsi per poter affrontare il mercato globale con nuovi strumenti più adatti. Quello che serve, inoltre, è uno stimolo al *marketing*, promuovendo le vendite oltre i confini tradizionali e favorendo soprattutto le esportazioni. È vero che nel passaggio cadono le garanzie e le tutele, ma è anche vero che per le imprese produttrici e commerciali di servizi si possono aprire nuovi mercati se riescono ad attrezzarsi adeguatamente. L'Italia deve essere più competitiva sul mercato internazionale. Le piccole e medie imprese rappresentano infatti la spina dorsale della nostra economia e inoltre nel settore commerciale garantiscono anche la distribuzione che è funzione sociale nei piccoli centri, un servizio di vicinato che deve essere garantito anche in futuro, soprattutto a favore delle persone anziane. Siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta. Auspichiamo però che il Governo tenga conto delle difficoltà di questo delicato passaggio, sviluppando un programma per le piccole e medie imprese. Condividendo le linee ed i princìpi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le autonomie a questo provvedimento e la nostra fiducia al Governo.

Presidente, una volta il benaltrismo era una categoria utilizzata dalla sinistra per motivare il fatto che le riforme non erano mai sufficienti; ora ci vuole ben altro, è un'espressione utilizzata dalla destra, per opporsi a provvedimenti, anche minimi, che vanno nella direzione di aprire i mercati, di creare più concorrenza nei mercati. Ad esempio, bisogna intervenire non con queste misure minime, ma sull'energia, sul gas, sui servizi pubblici locali. locali. È facile da parte nostra ricordare che, in cinque anni di Governo, la destra non ha fatto assolutamente nulla su questi settori, cioè sull'energia e sul gas in particolare. Anzi, la destra nei cinque anni precedenti ha bloccato l'inizio delle riforme che nella XIII legislatura i Governi di centro-sinistra avevano iniziato a realizzare.

detto - ma serve soprattutto a garantire trasparenza sui costi dei servizi per dare la possibilità agli utenti, eventualmente lo volessero, di cambiare operatore, se ritengono che il prezzo sia troppo alto.

che non trovano la possibilità di intraprendere e di realizzare iniziative nel mercato del lavoro, perché ci sono meccanismi che bloccano la possibilità di intrapresa, dei meccanismi chiusi che invece devono essere aperti. Inoltre, riteniamo che occorra garantire un servizio più ampio e competitivo nei confronti di tutti gli utenti. Infine, la questione forse più spinosa, sulla quale si è discusso, riguarda la revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità.

dicendo che bisogna avere mercati regolati, che bisogna garantire i mercati e che la concorrenza fa bene al mercato e ai consumatori; quando poi si

è la seguente: funziona veramente un mercato in cui si assegna la progettazione e la realizzazione delle opere senza gara pubblica?

I progetti in corso di realizzazione saranno completati; quindi, non c'è alcun rinvio. Per gli altri progetti, si farà la gara perché chi vince una gara ha tutto l'interesse a fare in fretta e a fare bene, mentre chi ha una concessione tende ad andare lento.

Colleghi, il *general contractor* ha prodotto danni all'erario, ha allungato i tempi e non ci sono stati i controlli che il pubblico doveva esercitare. Alta velocità Torino-Napoli, la spesa fissata dai contratti nel 1991 era di 5 miliardi di euro circa. Nel 2003, la spesa è aumentata a 23 miliardi di euro: il 410 per cento in più. Questo ha generato il *general contractor*; quindi, noi stiamo lavorando per creare più concorrenza, più trasparenza, più servizi, per cercare di far risparmiare i consumatori. Certo, eravamo aperti al confronto, ma c'è stata - ritengo - un'opposizione pregiudiziale. Ne prendiamo atto: vuol dire che c'è qualcuno in questo Paese che difende le corporazioni, i privilegi delle banche e delle assicurazioni, che preferisce assegnare gli appalti attraverso la trattativa privata. Questo è ciò di cui dobbiamo prendere atto. prendiamo atto, ma andiamo avanti. Il nostro voto sulla fiducia sarà un voto positivo per stimolare il Governo a proseguire su questa strada. L'opposizione ha parlato di Senato svuotato e la colpa ovviamente è del Governo che pone la fiducia. Io voglio solo ricordare che questo provvedimento è entrato alla Camera il 1° febbraio 2007

agli interessi degli utenti, della gente normale. Se farà questo, non solo avrà la fiducia del Parlamento ma anche del Paese. Noi siamo certi che questa sia la strada giusta. *(Applausi

per l'ennesima volta ci troviamo a votare una questione di fiducia posta dal Governo.

L'ho notato con piacere e aspettavo con ansia la sua replica alle domande più importanti e più incisive che sono state poi poste da tutti

alla semplificazione delle iscrizioni per via telematica, che sono state rimandate comunque a dopo il 15 maggio e che vedono le camere di commercio non ancora pronte ad attuarle. Ci spieghi, speravamo che ce le spiegasse spiegasse queste cose. Abbiamo chiesto anche con insistenza il perché pochezza e dell'impossibilità di discutere di norme che riteniamo importanti, sappiamo essere importanti, ma che nulla hanno a che vedere l'una con l'altra. Nulla hanno a che vedere la scuola con il decreto riguardante la tutela dei consumatori, tanto meno con la TAV, cui accennerò dopo. La decretazione d'urgenza, hanno detto, è stata colpa delle opposizioni portate avanti alla Camera. Sono andato ad esaminarmi i numeri per vedere come si è lavorato alla Camera e come questo Governo ha chiesto di lavorare. Portate pazienza se ve li elenco un attimo.

si arriva al giorno 22 marzo, ultimo giorno in Commissione. Sono 19 giorni di lavoro e in questo periodo la somma dei tempi delle sedute è pari a 23 ore e 35 minuti: si è quindi lavorato un'ora e mezza a seduta.

Se non ricordo male, nel frattempo vi è stata una profonda crisi di questo Governo e tutta l'attività parlamentare si è dovuta fermare per risolvere i problemi all'interno della maggioranza. Pertanto, amici miei, non diamo la colpa alla giusta e doverosa opposizione delle minoranze. Non diamo la colpa. Signor Ministro, ho visto che prendeva nota anche su altri punti importanti, ma punti importanti, ma non ho avuto risposte quando ho toccato il problema dell'ISVAP, non ho avuto risposte quando le ho chiesto delle

che sostenga che discutere di barbieri sia poca cosa. Non credo che la stampa anglosassone si venga ad interessare dei barbieri italiani, porti pazienza. *(Applausi dal Gruppo LNP)*. Con questo non diciamo che non si doveva fare la liberalizzazione, ma citare la stampa anglosassone, amici miei, in questo caso

che speravamo fosse veramente il dialogo auspicato e sollecitato, insieme a quelle risoluzioni *bipartisan* che continuate a predicare ma che poi in realtà non volete, amici miei. Questa è la reale verità. Per Per entrare nel merito, colleghi, signor Presidente, sulla liberalizzazione dei servizi assicurativi abbiamo chiesto espressamente

è l'ente che provvede alle liquidazioni coatte, a liquidazioni in piedi da quasi vent'anni. Signor Ministro e signori del Governo, queste sono le cose a tutela dei consumatori su cui si dovrebbe intervenire!

riguardanti il blocco delle opere pubbliche. A parte il fatto che quando sento che i colleghi

fare», sul blocco delle opere pubbliche, amici, bisognava fare una riflessione, ecco perché non poteva essere inserito in questo provvedimento. Bisognava veramente fare una riflessione che ci portasse che ci portasse a ragionare sul reale prezzo da pagare per bloccare queste opere pubbliche. Come viene vista la cosa dal punto di vista degli investitori esteri? Voi sapete che gli investimenti dall'estero in questo Paese continuano a calare. Non domandatevi il perché: il perché sta in questi comportamenti. Che fiducia può avere un investitore estero in un Paese come il nostro che revoca una concessione di diritto acquisito? Questo non è più lo Stato del diritto; neanche nei Paesi sottosviluppati, neanche nei Paesi dell'America Latina succedono queste cose.

Presidente, concludo. È inutile che vi riempite la bocca con il sostegno alle piccole imprese. Le piccole imprese si trovano soprattutto in Padania, dove voi avete cancellato quelle opere pubbliche programmate e finanziate nel 1991, che non hanno ancora avuto luogo; ma non è questo il sistema per accelerare il loro sviluppo e la loro esecuzione.

non appartengo alla maggioranza governativa, né intendo iscrivermi. Sono convinto, però, della bontà di queste norme e so anche anche apprezzare il fatto che il ministro Bersani è stato presente a tutta la discussione e ha dato ieri delle risposte molto esaurienti in un'Aula che non era molto affollata. Per questi motivi voterò a favore, nonostante sia voto di fiducia.

Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, sul decreto-legge n. 7 del 2007, la cosiddetta seconda lenzuolata di liberalizzazioni proposta dal ministro Bersani, si possono in parte ripetere considerazioni svolte sul primo decreto Bersani del luglio scorso. Anche in questo caso, infatti, si adotta il termine «liberalizzazioni» con molta disinvoltura, salvo poi scoprire che le misure adottate sono di spessore molto modesto e del tutto insufficienti rispetto all'obiettivo preannunciato. Quindi anche questa volta siamo costretti a far notare al ministro Bersani quanto tutto ciò appaia riduttivo ed insufficiente rispetto ai reali bisogni dei cittadini. Non è certo di queste liberalizzazioni, del tutto marginali e insignificanti, che il Paese ha bisogno, nonostante si insista nel voler far credere all'opinione pubblica il contrario. Le vere liberalizzazioni, quelle in grado di incidere sugli assetti del mercato, aprendo la porta alla concorrenza laddove ci sono delle situazioni di monopolio od oligopolio, e di avvantaggiare concretamente i cittadini, sono di tutt'altra natura ed investono ed investono settori quali i servizi pubblici locali, il trasporto e la pubblica amministrazione. E appare davvero contraddittorio e sospetto che il disegno di legge Lanzillotta, relativo proprio alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, stenti ad andare avanti in Commissione affari costituzionali al Senato, mentre le misure contenute nel provvedimento in esame siano considerate, solo queste, estremamente urgenti. Le vere liberalizzazioni rimangono, quindi, insabbiate e sono annacquate con emendamenti che ne diminuiscono sensibilmente la portata, mentre le finte liberalizzazioni godono di una corsia preferenziale: vorrei che il Governo ci spiegasse quale criterio determina questo tipo di scelte, perché a noi risulta davvero oscuro a capirsi. L'utilizzo, ancora una volta, della decretazione d'urgenza, infatti, è assolutamente ingiustificato, visti i contenuti, e comunque non adeguato ad affrontare temi da voi ritenuti così importanti, su cui dovrebbe esserci un dibattito ampio e costruttivo in Parlamento, con la possibilità anche per l'opposizione di esporre le proprie posizioni e apportare il proprio contributo. Ma, come per il primo decreto Bersani, temiamo che anche in questo caso l'uso del decreto-legge nasconda ben altre finalità. Lì si trattava del *blitz* del vice ministro Visco in materia fiscale, qui si interviene sulla TAV e sulla scuola, materie che francamente, neanche con il più grande sforzo di fantasia, possono essere ricondotte alle liberalizzazioni. Ma ancor più grave è il fatto che l'esame del provvedimento in Parlamento sia stato ulteriormente ristretto con l'apposizione della questione di fiducia non solo alla Camera, ma anche al Senato. Infatti, se l'uso del decreto-legge riduce di molto la possibilità di dibattito e di modifica del provvedimento, l'apposizione della fiducia la elimina del tutto. Il nostro partito ha posto anche al Capo dello Stato il problema istituzionale e ieri il nostro Capogruppo lo ha ripetuto alla Conferenza dei Capigruppo del Senato. E che si dica che la richiesta di fiducia si è resa necessaria a causa del comportamento irresponsabile dell'opposizione mi sembra davvero una mistificazione della realtà. Le proposte dell'UDC erano serie e miravano a migliorare il testo, tant'è vero che alcune di esse, in materia di banche e assicurazioni, sono state recepite nel corso dell'esame alla Camera. La verità, come in altre occasioni, è che l'accusa di ostruzionismo all'opposizione è solo il pretesto per nascondere la paura di non reggere la prova del confronto parlamentare, soprattutto qui in Senato che si trova ancora una volta nell'impossibilità di esaminare il provvedimento e di apportare contributi migliorativi. E che questo Governo non sia in grado di gestire la sua maggioranza è sotto gli occhi di tutti: e non è solo la politica estera a determinare le distanze tra le diverse componenti, cosa di per sé già molto grave, perché non c'è un solo argomento su cui ci sia una posizione convergente. Una delle misure contenute nel decreto riguarda, per esempio, proprio la TAV su cui pesa fortemente la contrarietà della sinistra radicale. E per risolvere la situazione si è pensato bene di congelarla, revocando le concessioni già rilasciate nel 1992. Come questo abbia a che fare con le liberalizzazioni e come possa rispondere all'interesse del Paese è davvero difficile capirlo, visto che non si fa altro che rallentare la realizzazione di un progetto infrastrutturale, relativo alle reti di trasporto europee, di fondamentale importanza, senza considerare il contenzioso che nascerà da questa norma ed i relativi costi. *(Applausi dal Gruppo* *UDC).* Non è cancellando gli impegni contrattuali dall'alto che si sostiene la crescita del Paese: l'effetto che si produce è solo la perdita di credibilità ed il sospetto che ciò venga fatto per favorire alcune imprese, ripeto, alcune imprese, senza considerare che si andrà a penalizzare fortemente il fattore occupazionale, se sono vere le notizie di questi giorni sulla soppressione di circa 6.000 posti di lavoro. Non si comprende neanche cosa c'entri l'articolo 13 sulla formazione professionale e quali siano i requisiti di urgenza per trattare tale materia in un decreto‑legge. Il vero fine è demolire un pezzo alla volta le riforme attuate nella precedente legislatura, non proponendo dei progetti alternativi ed organici, ma con dei veri e propri *blitz*. Ma la scuola non è un tema da trattare con leggerezza e superficialità come fa questo Governo, liquidandolo in un provvedimento d'urgenza. L'intervento del Governo, infatti, riporta al passato la formazione professionale, con l'abolizione del liceo tecnologico e di quello economico, e solo grazie agli emendamenti dell'opposizione è rimasto il riconoscimento della pari dignità del sistema dell'istruzione e formazione professionale. Il criterio guida della politica del Governo non può essere il *furor* ideologico, con conseguente smantellamento sistematico delle riforme del centro‑destra, a prescindere dal contenuto. Bisogna avere l'onestà di riconoscere quanto di buono c'è nelle riforme attuate dal precedente Governo, e semmai migliorarle, non cancellarle. Se si continua ostinatamente a sostenere che la riforma della scuola non ha innovato il sistema dell'istruzione, che la legge Biagi ha portato solo precarietà, che la riforma delle pensioni è stata insufficiente, non si fa certo il bene del Paese. Tutte queste riforme hanno il merito di avere affrontato, in un ampio e lungo dibattito parlamentare nella precedente legislatura, temi fondamentali in modo sistematico e serio. Ma vorrei esprimere tutte le nostre perplessità anche sulle pretese liberalizzazioni contenute nel decreto, che si riducono nella sostanza a ben poca cosa. Piuttosto, le definirei delle vere e proprie penalizzazioni, ripeto, penalizzazioni, poiché si continua a procedere con il metodo della liberalizzazione selettiva, scegliendo alcune categorie da colpire, come se da esse dipendesse l'andamento dell'economia italiana. Non mi sembra che gli acconciatori, i panificatori, le guide turistiche e i facchini rappresentino settori su cui era necessario intervenire d'urgenza, e non credo che i consumatori avranno particolari benefici dalla liberalizzazione di queste attività. Non è un intervento liberalizzatore neanche la soppressione delle ricariche telefoniche, di cui, tra l'altro, non si valutano bene le conseguenze rispetto alla possibilità che le compagnie aumentino i costi del traffico telefonico, come è presumibile che avvenga, scaricando sui consumatori i mancati introiti delle ricariche. Altro che vantaggi per i consumatori! In tale ambito, come da molti sottolineato, sarebbe stato meglio non intervenire normativamente, ma lasciare spazio ai poteri regolativi dell'Autorità delle telecomunicazioni, che già si stava occupando della materia. Un reale beneficio per i consumatori - e su ciò ha convenuto anche la maggioranza in Commissione - sarebbe invece derivato, come richiesto dall'opposizione, dall'abolizione delle tasse di concessione governative, il cui peso, in termini percentuali, è ben maggiore delle ricariche. E ancora, con la norma sull'eliminazione della penale per l'estinzione anticipata dei mutui non si opera l'apertura alla concorrenza di un mercato, ma si interviene in materia di contratti tra privati, mentre sarebbe stato meglio rafforzare i poteri di controllo e di intervento della Banca d'Italia sulla trasparenza del mercato bancario e sull'effettiva possibilità per i consumatori di confrontare i prodotti offerti. Anche in tal caso non si può escludere un effetto dannoso per i consumatori dovuto all'innalzamento dei tassi di interesse. In parte apprezzabili e condivisibili sono le misure di semplificazione amministrativa per le imprese: ma anche qui si tratta di vedere come lo *slogan* «impresa in un giorno» potrà tradursi in realtà di fronte alle note resistenze e lentezze dell'apparato burocratico. In conclusione, a questo si riducono le piccole misure? A questo proposito, signor Ministro, forse ha ragione lei, non sono piccole, ma sono sicuramente insignificanti le misure che si vogliono spacciare per liberalizzazioni, e che permetterebbero di agganciare la ripresa economica in atto nel Paese. È per questo che noi dell'UDC siamo convinti che le scelte strategiche da operare siano ben altre: cioè attuare liberalizzazioni vere, che significhino apertura dei mercati alla concorrenza, e che riguardino prima di tutto settori nevralgici dell'economia e non piccole categorie marginali e del tutto ininfluenti; occorre, inoltre, avviare subito un dibattito serio sulle pensioni; infine, è necessario alleggerire il carico fiscale per le famiglie utilizzando in parte le risorse provenienti dall'extra-gettito fiscale, il cosiddetto tesoretto. Sono queste, e non le inutili cosiddette lenzuolate, le priorità dell'agenda politica per l'UDC e su questi temi siamo pronti e disponibili ad un dibattito serio e costruttivo, finalizzato ad adottare le politiche necessarie per sostenere l'attuale favorevole congiuntura economica a promuovere concretamente il benessere dei consumatori e delle famiglie, a patto, però, che non ci siano pregiudizi o barricate ideologiche da parte di una maggioranza preoccupata solo di sopravvivere sullo scarto di un paio di voti. Ciò che sicuramente non accettiamo è di essere il capro espiatorio di questa maggioranza così divisa al suo interno, e quindi debole e litigiosa. Sono tutte queste le motivazioni

Signor Presidente, il decreto che ci apprestiamo a convertire in legge, e per il quale Rifondazione Comunista-Sinistra Europea voterà convintamente la fiducia al Governo, affronta temi sensibili per tutti i cittadini, ma particolarmente per quelli che con difficoltà arrivano a fine mese, per quelli che - come ci dice oggi il rapporto EURISPES - hanno visto i loro redditi abbassarsi sempre di più in rapporto ad un'inflazione che invece è cresciuta. Riguarda le ricariche telefoniche, la libertà di cambiare gli operatori telefonici, televisivi e di Internet, l'informazione sui prezzi dei carburanti, la leggibilità e trasparenza delle tariffe aeree, l'obbligatorietà dell'apposizione della data di scadenza dei prodotti alimentari, la concorrenza nei servizi assicurativi, la semplificazione nella cancellazione delle ipoteche immobiliari, l'estinzione anticipata dei mutui senza oneri e penali, la portabilità dei mutui, la tutela degli utenti di banche e assicurazioni da spese ingiustificate; e poi la scuola, la revoca delle concessioni la semplificazione amministrativa, la liberalizzazione nell'accesso in alcune professioni. «Molto rumore per nulla», ha detto l'opposizione, cioè ha minimizzato trattandosi di un provvedimento, per così dire, minore, che non tocca le liberalizzazioni importanti di quei settori, energia, gas, ferrovie e poste, attraverso i quali si modificano gli assetti fondamentali dell'economia del Paese. Si è detto con accenti spesso anche derisori che questo provvedimento riguarda cose minute: attenzione però che la derisione destinata nella polemica politica alle norme contenute nel provvedimento non si riverberi sui concretissimi affanni di persone reali, per cui 5 euro su ogni ricarica telefonica, un minor costo dell'assicurazione o una minore soggezione verso la banca sono benefìci che contribuiscono a migliorare la vita quotidiana; tendono ad un certo riequilibrio della spropositata asimmetria di potere tra utente e i soggetti economici e finanziari; ancora mutano, positivamente il rapporto fra Stato e cittadini. Certo, sono piccoli passi, ma nella giusta direzione della tutela dei diritti dei cittadini e delle cittadine, della mitigazione delle vessazioni, dei soprusi, del potere delle istituzioni più forti nella nostra società. Non si tratta di esaltare oltre misura questo provvedimento quanto di porre l'attenzione su una attitudine per noi fondamentale: quella di trasformare la frustrazione, l'impotenza e la solitudine di ogni cittadino utente di fronte a regole incomprensibili e gabelle ingiuste in fiducia nello Stato, inteso come soggetto capace di rappresentare il bene comune e gli interessi generali e sociali; di essere permeabile alle richieste di quei ceti popolari sempre così poco rappresentati, la cui voce arriva solo in modo intermittente (forse perché essi non dispongono di uffici per i rapporti con il Parlamento) e per i quali le opportunità di risparmio sono vitali nella percezione di una maggior sicurezza nella conduzione della propria vita. Di questo Stato c'è bisogno, perché la difesa degli interessi generali non è la somma caotica di tanti particolarismi, ma qualcosa di più alto, come ci insegna la Costituzione italiana. Non è certo questo a cui ci ha abituati il Governo precedente, segnato dall'uso privato della cosa pubblica, dagli interessi e dalla voracità di pochi elevati a misura dello sviluppo del Paese, che negli anni della sua legislatura non è riuscito a mettere in campo nemmeno uno dei provvedimenti su cui oggi votiamo su cui oggi votiamo la fiducia e che ancora nel dibattito odierno li irride; provvedimenti che riguardano anche il tema dello sviluppo economico del Paese, dello svecchiamento di alcune sue strutture, nel senso di una capacità competitiva fondata sulla qualità e il rinnovamento, piuttosto che su rendite di posizione e tutele corporative. Con questa attitudine, che apprezziamo, con questo medesimo atteggiamento auspichiamo saranno affrontate le questioni centrali per una pienezza della cittadinanza: la condizione di lavoratori e lavoratrici precari, la condizione dei pensionati, dei disoccupati e dei migranti, cioè i temi dell'equità, della redistribuzione e del risarcimento sociale. Nel dibattito si è ironizzato sulla effettiva efficacia della riduzione dei prezzi prevista da alcune norme sottolineando come esse saranno facilmente raggirate sia dagli operatori della telefonia mobile, sia dal sistema finanziario e che, quindi, non cambierà nulla: non diminuiranno i costi della ricarica e non compreremo prodotti assicurativi più convenienti. Può essere che ciò accada perché, in effetti, il mercato non è il luogo dell'equità. La pressione concorrenziale da sola non è sufficiente garanzia per gli utenti; la libertà del consumatore è spesso solo quella di scegliere da chi essere abbindolato perché il consumatore, in quanto tale, non è neanche libero di scegliere se consumare o no. Noi questo lo sappiamo. Che lo affermino anche i vessilliferi delle virtù del libero mercato ci colpisce come una nota stonata che dovrebbe consigliarli a cambiare musica. Ma poiché noi ne siamo consapevoli, tentiamo di ridurre, anche con questa legge, i danni prodotti dal sistema e, soprattutto, siamo determinati a sottrarre dal mercato e dalle sue pretese beni come l'acqua, ma l'ambiente tutto, la salute, l'istruzione, che sono di tutti e di ognuno e tali devono rimanere. Già molto si è detto nel merito del provvedimento, mi soffermo brevemente su alcuni aspetti per un ripasso veloce. Per quel che riguarda il costo improprio delle ricariche telefoniche, voglio ricordare che gli utilizzatori della ricarica sono soprattutto i ragazzi, i giovani e i migranti e che, quindi, quel balzello gravava soprattutto sulle loro spalle e che solo nel nostro Paese la ricarica era gravata da un costo supplementare su cui la Commissione europea ci ha chiesto di fare chiarezza. Ricordo ancora che il Governo ha recepito la forte sollecitazione che è arrivata dalla petizione firmata da migliaia di cittadini e che di questo dobbiamo ringraziare - voglio ricordarlo - Andrea D'Ambra, il giovane che non si è accontentato e che ha avuto fiducia nella possibilità di cambiare. Sappiamo che nel nostro Paese l'80 per cento circa della popolazione vive in una casa di proprietà, a ciò sospinta dalla carenza cronica di interventi, dall'offerta di edilizia pubblica e da un mercato degli affitti insostenibile: come non cogliere il sollievo di quanti, costretti a scegliere se far studiare i figli o vivere con un po' di stabilità, casa hanno acceso un muto e sono ora sgravati dal costo dell'ipoteca e da quello dell'estinzione del mutuo? Come non apprezzare che banche, istituti di credito, assicurazioni non possano più addebitare le spese per l'estratto conto o gli avvisi di pagamento? Che le società di assicurazione - che quanti posseggono un veicolo a motore sono obbligati a stipulare - debbano applicare contratti più favorevoli all'assicurato non potendo imporre, ad esempio, il pagamento del premio per la classe più alta a chi cessi per un periodo il contratto e poi lo riattivi? Regole arbitrarie, premianti per le assicurazioni, che non hanno un fondamento oggettivo. All'articolo 2 sono stabilite misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza che devono rimandare ad un ruolo propositivo, propulsivo e progettuale delle amministrazioni locali. Le misure prevedono l'accelerazione dei tempi per la nascita di nuove imprese centrata sulla semplificazione amministrativa e sull'implementazione dell'impiego di mezzi telematici, cioè, maggiore efficienza degli *iter* procedurali, ma in un contesto di regole e di controlli certi, a garanzia del territorio e della popolazione. alcune attività economiche, quali autoscuole, parrucchieri e parrucchiere ed estetiste, attività di facchinaggio, pulizia e disinfezione sono deregolamentate al fine di migliorare la qualità del servizio reso, ma anche per offrire opportunità di accesso al lavoro e di intraprendere attività autonome. Sappiamo quanta della formazione professionale delle giovani donne sia ancora concentrata nei settori delle acconciature e delle cure estetiche: consentire loro uno sbocco lavorativo è importante, ma non si può prescindere da interventi per assicurare il più possibile la solidità di queste attività. la liberalizzazione dell'attività di accompagnatore e di guida turistica ha il fine di offrire opportunità di lavoro a neolaureati disoccupati in un ambito rilevante dell'economia del Paese legato al turismo e all'accoglienza dei turisti. A mitigare la preoccupazione che la liberalizzazione comporti uno scadimento della qualità delle competenze degli operatori, la Camera ha introdotto la previsione che le Regioni possano utilizzare sistemi di accreditamento, cioè operare per la qualità e la competenza degli operatori del settore definendo le caratteristiche e le condizioni migliori di sviluppo dell'attività per quel determinato territorio, anche in ordine alla tipologia del rapporto di lavoro. lavoro. Il ruolo delle amministrazioni locali, quindi, può essere propulsivo, se lo si concepisce come promotore, orientatore, formatore, accompagnatore, incubatore di attività economiche insieme agli attori dei processi economici. Non è solo farraginoso apparato burocratico, quindi, ma dinamico attore del territorio a patto di dargliene i mezzi, le risorse e la cultura. Sulla scuola è già stato sottolineato come il merito principale del provvedimento, così come è stato rielaborato dalla Commissione competente della Camera, è stabilire che il sistema di istruzione secondaria è un sistema unico nel quale si valorizza l'area dell'istruzione tecnico-professionale. Perplessità permangono invece sul tema delle donazioni alle scuole pubbliche e paritarie: riteniamo che il sistema di finanziamento debba avvalersi della fiscalità generale e che le donazioni possano produrre forti disparità tra scuole, che dovranno essere recuperate dal fondo di perequazione. La revoca delle concessioni per la costruzione delle linee di TAV - l'ha specificato ancora ieri il ministro Bersani - non è, purtroppo, dal nostro punto di vista, il ripensamento complessivo sull'avventura delle infrastrutture concepite senza pianificazione e senza rispetto per il territorio, con costi dalle tre alle cinque volte comparativamente superiori a quanto avviene in altri Paesi europei: è però una misura di autodifesa messa in atto dallo Stato per la trasparenza e la riduzione dei costi, per l'applicazione della normativa europea sull'affidamento tramite gara e per questo l'apprezziamo. Ben venga, quindi, e vediamo di fare di necessità virtù, cioè di stabilire le priorità delle opere, a partire da un piano dei trasporti complessivo. Cito, infine, l'articolo 11 che prevede misure per il mercato del gas, per determinare la concessione di aliquote del prodotto dovute dai titolari delle concessioni allo Stato: è una misura importante, di cui discuteremo nel prossimo futuro,

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, questa è la diciassettesima fiducia che il Governo Prodi pone. Al di là del fatto che chi crede alla Cabala e ai numeri soprattutto da parte della maggioranza farebbe meglio a fare i debiti scongiuri, visto il numero, siamo alla diciassettesima fiducia nel corso di meno di un anno di questo Governo, il che significa l'esproprio delle Camere e del dibattito parlamentare. Per giunta, un argomento come questo, molto delicato,

Quindi, non è vero che siete arrivati alla fiducia solo ed esclusivamente perché vi è stato l'ostruzionismo dell'opposizione alla Camera: siete arrivati alla fiducia al Senato perché questa è una fiducia politica. Con i numeri ballerini che avete in quest'Aula, temevate che questo provvedimento venisse cambiato in maniera pesante, che qualche emendamento dell'opposizione fosse approvato e che, quindi, snaturasse questo provvedimento che così faticosamente avete costruito. Il ministro Chiti ha dichiarato ieri che non si aspettava di dover contrastare in Aula l'opposizione del centro-destra su un decreto concernente le liberalizzazioni. Ma questo, signor Presidente, signori del Governo, colleghi, non è un decreto-legge sulle liberalizzazioni; semmai è un provvedimento sulle deregolamentazioni. Deregolamentazioni di alcune categorie che sono assolutamente e politicamente lontane dal Governo e dalla sua maggioranza. Liberalizzazioni non concordate con le categorie, con le associazioni, e concordate tutt'al più con qualche associazione di consumatori. E queste ultime, come è noto, al di là di qualche avvocato, nel maggior numero dei casi rappresentano solo se stesse.

solito dire io - dei poveracci, di chi si è aperto una partita IVA, di chi ha cominciato a lavorare in proprio, di chi ha impegnato il proprio denaro: le liberalizzazioni delle autoscuole, delle guide turistiche, delle assicurazioni,

con il rischio che queste norme creino monopoli che vadano a procurare nuova disoccupazione. Non soltanto avete

rispetto al monomandatario, signori che mi ascoltate, pensate sia a favore dell'agente della compagnia di assicurazione o dei clienti? Secondo voi, l'agente plurimandatario

che gli fornisce una maggiore provvigione sulle vendite? Cominciamo a ragionare su questi aspetti e se queste norme vanno davvero incontro al cittadino oppure rispondono solo ed esclusivamente ad alcune

che la questura di Roma abbia impedito alle guide turistiche di venire a manifestare davanti al Senato per portare avanti le loro rivendicazioni.

collega Valditara. Consentitemi però di parlare della TAV, della norma di cancellazione delle concessioni dell'alta velocità.

poiché sta mimetizzando, all'interno di un provvedimento inutile, un suo sfogo personale nei confronti del passato Governo che aveva riportato nella legittimità un atto che proprio lo stesso ministro Bersani nel 2000 aveva portato avanti azzerando i contratti avallati dal Consiglio di Stato. Gli italiani devono sapere

Il ministro Bersani, in modo irreversibile, sta ponendo fine alla realizzazione di opere essenziali per il Paese e per l'Europa, in quanto si tratta di opere ubicate su corridoi transeuropei per le quali questo Paese non potrà più disporre di risorse dell'Unione Europea. Ma è ancora più grave che il ministro Bersani stia realizzando un vero e misurabile conflitto di interessi regalando ancora una volta al mondo delle cooperative un possibile ed enorme teatro di convenienze, mimetizzando la sua azione come azione ricca di trasparenza. Mi chiedo, infatti, quale possa essere l'impresa straniera che verrà a partecipare a gare su tali lavori senza essere costretta ad allearsi, e - come si dice nel gergo della sinistra - a consorziarsi per acquisire tali lavori. Come già sta avvenendo su una serie di eventi, quali quelli che le Ferrovie dello Stato e l'ANAS hanno già verificato in merito all'assenza di risorse della finanziaria derivanti dal TFR, i cittadini di questo Paese capiranno subito la falsità del provvedimento ed il danno irreversibile che lo stesso produce. Ministro, questo non glielo perdoneranno e al momento del voto sapranno chi è stato il diretto responsabile di questa crisi di crescita, di questa falsa azione di liberalizzazione. Il ministro Bersani non sta fermando solo un treno in corsa (perderemo infatti almeno due anni per una simile folle iniziativa), ma sta fermando il treno dello sviluppo. Voglio solo ricordare che mentre noi discutiamo e ci affanniamo per bloccare interventi sulla rete dell'Alta velocità, l'Europa realizza contestualmente il triplo delle reti che noi stiamo bloccando. Signor Presidente, colleghi, il no di Alleanza Nazionale è un no duplice: no a questo provvedimento e no alla fiducia a questo Governo che sta penalizzando l'Italia, la sua economia e i suoi cittadini.

colleghe e colleghi, anticipo subito che Forza Italia esprimerà un convinto voto contrario al Governo per la fiducia posta sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 7. Siamo contrari al provvedimento per tanti motivi. Innanzitutto il decreto legge viola le condizioni previste dall'articolo 77, della Costituzione per l'uso da parte del Governo di tale delicato strumento legislativo: dove sono nel provvedimento i casi straordinari di necessità e di urgenza che giustificano il decreto-legge? All'articolo 13, si arriva al colmo di effettuare per decreto legge la riforma dell'istruzione tecnico-professionale! Purtroppo, questo Governo ricorre ormai sistematicamente a questo grave abuso costituzionale, perché realizza così una sostanziale limitazione dell'azione di controllo legislativo del Parlamento, dove al Senato la maggioranza è piuttosto risicata. A voi, cari colleghi, giudicare quanto questo comportamento sia coerente con l'impegno a valorizzare la centralità del Parlamento, un anno fa sbandierato con enfasi nelle pagine del programma dell'Unione. Dobbiamo rilevare in secondo luogo che al Senato i tempi limitatissimi a disposizione per il provvedimento (ridotti a cinque concitati giorni) ne hanno impedito un serio esame. È un'altra grave lesione della Costituzione, là dove all'articolo 70, è previsto che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente da Camera e Senato in piena eguaglianza. Ad esaminare il provvedimento è stata praticamente solo la Camera, che ha usufruito del 90 per cento del tempo disponibile, signor Presidente, tra l'altro buttando via 16 giorni senza far nulla. Di fatto siamo al monocameralismo. Di tale malfunzionamento qualcuno del Governo o della maggioranza è colpevole o per incapacità gestionale o, peggio, per perversa strategia. Il ministro Bersani con un grande *battage* mediatico ha presentato il decreto legge all'opinione pubblica come fondamentale contributo alla liberalizzazione del Paese. Ad un esame obiettivo tale presentazione risulta invece mistificante. Le liberalizzazioni effettivamente operate sono di importanza modesta: i parrucchieri e gli estetisti potranno lavorare anche il lunedì; avremo informazioni migliori sui prezzi del carburante in autostrada; gli adempimenti per attivare un'impresa di pulizie saranno ridotti al minimo; alle tariffe aeree sarà assicurata una miglior trasparenza, ma permane intatta la gigantesca montagna di lacci e lacciuoli che vincola in mille modi i cittadini italiani, con un enorme cumulo di leggi, decreti e regolamenti, spesso ambigui e contraddittori, con il groviglio di burocrazie centrali, regionali, provinciali e comunali, con i sistematici ritardi nelle decisioni della pubblica amministrazione, con le centinaia di imposte e tasse, eccetera. La liberalizzazione è un'esigenza primaria urgentissima per la modernizzazione della società italiana. Ad essa il contributo di questa «lenzuolata» è davvero minimo. Assieme a poche mini-liberalizzazioni, utilizzate come paravento mediatico, il provvedimento al nostro esame contiene purtroppo alcune disposizioni ispirate da ideologie stataliste e dirigiste che ledono fondamentali libertà, vitali per il funzionamento della nostra società. Mi soffermerò in particolare sulle disposizioni di cui agli articoli 1, 5 e 13. Al comma 1 dell'articolo 1 viene introdotto il divieto per gli operatori di telefonia dell'applicazione di costi fissi per la ricarica di carte prepagate. Agli operatori vengono lasciati appena 30 giorni per adeguare l'offerta commerciale alla platea degli utenti (che sono decine e decine di milioni). I 30 giorni sono stati fatti decorrere non già dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto-legge, come sarebbe stato necessario per rispetto del Parlamento, ma dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, precostituendo così condizioni da cui è impossibile tornare indietro. La tecnica è quella del fatto compiuto. La disposizione, comportando per le imprese del settore una minor entrata complessiva di circa 2 miliardi di euro, sballa i piani industriali e distorce l'assetto concorrenziale del settore, dato che grava su imprese con assai diversa capacità di tenuta finanziaria. Va inoltre notato che nel settore opera con piena competenza l'Autorità garante per le comunicazioni, che in effetti stava già studiando un provvedimento del genere. Questo intervento a gamba tesa del Governo, in un delicato settore del mercato risulta a tutti gli effetti privo di seria motivazione. L'evidente obiettivo risulta la demagogica cattura del consenso che segue all'atto della cancellazione di una voce di costo nella bolletta telefonica.

elimina la possibilità di clausole contrattuali di distribuzione in esclusiva di polizze assicurative riguardanti i rami danni. Presentata dal Governo come misura di liberalizzazione, è in realtà l'esatto contrario. Fino alla data di introduzione del decreto-legge non era infatti presente nella nostra legislazione nessun obbligo di distribuzione in esclusiva. L'esclusiva rappresentava una delle varie modalità possibili nel mercato per la vendita dei prodotti assicurativi e si era affermata proprio per le sue superiori qualità. La copiosa letteratura scientifica in argomento dimostra con assoluta evidenza che le reti agenziali in esclusiva consentono di abbattere i costi medi della distribuzione e di offrire i prezzi più contenuti agli assicurati. E dimostra altresì che gli agenti plurimandatari tendono a proporre i prodotti per essi più remunerativi in termini di provvigione. Segnaliamo che tale divieto di esclusiva non esiste in alcun altro Paese dell'Unione Europea e viola la direttiva n. 2002 del 1992 della Comunità Europea, che contempla espressamente la possibilità di ricorrere allo strumento del mandato in esclusiva. La disposizione inoltre indebolisce il sistema assicurativo nazionale rispetto ai concorrenti stranieri, che potranno giovarsi, senza alcuna necessità di investimento, delle reti distributive costruite e finanziate fino ad oggi dalle imprese italiane, e vìola altresì il diritto comunitario della concorrenza e della libera circolazione dei servizi nella comunità. C'è da chiedersi cosa abbia mosso il Governo a questa dissennata disposizione, che non produrrà benefici per gli assicurati e sarà presto dichiarata nulla perché contraria alle regole comunitarie.

solo perché la cultura di questo Governo per le sue ascendenze ideologiche è incapace di accogliere le giuste esigenze dei comparti produttivi del Paese. Infine all'articolo 13 il provvedimento revoca le concessioni rilasciate dall'ente Ferrovie dello Stato alla TAV S.p.A. nel 1991 e nel 1992, relative alle tratte ad alta velocità ed alta capacità Milano-Verona , Verona-Padova e Milano-Genova e Milano-Genova ed estende gli effetti delle revoche a tutti i rapporti convenzionali con i contraenti generali da esse derivati. Il gravissimo atto, motivato da obiettivi di risparmio sui costi di tali opere (risparmi che un'attenta analisi dimostra assolutamente non realistici) avrà purtroppo come primo e certo effetto la paralisi per anni della realizzazione di queste fondamentali infrastrutture del Paese. Questo ritardo renderà inoltre molto più a rischio il finanziamento di miliardi di euro promesso dall'Unione Europea per tali opere che fanno parte del Corridoio 5 Lisbona-Kiev e del Corridoio n. 24 Rotterdam-Genova. Inoltre, il decreto-legge, prevedendo l'inevitabile insorgere di un contenzioso tra i contraenti generali e la Ferrovie dello Stato spa, stabilisce pesanti deroghe all'attuale normativa concernente gli indennizzi in caso di revoche da parte della Pubblica amministrazione aventi incidenza su rapporti negoziali. In questi casi, con effetto retroattivo, l'indennizzo verrà non solo parametrato esclusivamente al danno emergente (escludendo il lucro cessante), ma dovrà anche tener conto dell'eventuale conoscenza o addirittura addirittura "conoscibilità" da parte dei contraenti degli elementi determinanti la revoca. Siamo allo scardinamento di fondamentali regole giuridiche. Le disposizioni, evidentemente ispirate da una marcata concezione statalista, sono in contrasto con gli articoli 3, 41, 42, 77, 81 e 113 della nostra Costituzione. In particolare, la limitazione dell'indennizzo viola la pienezza di esercizio della funzione giurisdizionale, garantita dall'articolo 113. Questa nuova regolamentazione avrà tra l'altro l'effetto di minare la certezza del diritto nei rapporti dei privati con la pubblica amministrazione e potrà persino avere ricadute sulla valutazione del *rating* del nostro Paese effettuata dalle agenzie internazionali specializzate. Siamo agli antipodi rispetto a ciò che occorrerebbe fare per tener conto della dinamica del processo di globalizzazione. Riscontriamo anche qui una forma di arroganza incompatibile con lo spirito di servizio dei veri interessi del Paese, che questo Governo, come ogni Esecutivo, deve sempre avere per propria stella polare.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il decreto-legge che ci accingiamo ad approvare, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia esclusivamente per ragioni legate alla ristrettezza dei tempi rimasti a nostra disposizione per la sua conversione in legge, è fortemente atteso dai cittadini, dalle famiglie, dai consumatori e dalle imprese. Esso, infatti, unitamente ad altri provvedimenti all'esame del Parlamento, risponde all'esigenza di un più ampio sviluppo della nostra economia e di un più corretto e moderno funzionamento dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione alle imprese e da queste ultime al cittadino. fattori sono fortemente mancati nel corso degli ultimi anni e su di essi il precedente Governo ha ottenuto i risultati negativi che bene conosciamo e ammessi dallo stesso onorevole Berlusconi il quale, ancora poche settimane fa, ha riaffermato che il suo Governo non ha fatto le liberalizzazioni per via delle divisioni che vi erano nella sua coalizione. Il baricentro del provvedimento sta nella necessità tutelare il cittadino, di dare una spinta alla crescita economica del nostro sistema, utilizzando gli strumenti della concorrenza, del rispetto delle regole, della semplificazione amministrativa e dell'abbattimento delle barriere burocratiche.

che riprendono, in parte, segnalazioni provenienti dall'Unione Europea e dalle autorità di settore. Come si può giustificare, in tal senso, la contrarietà alla soppressione di un costo ingiusto come quello sulle ricariche dei cellulari e dei servizi Internet e *pay* TV o a quella dei costi relativi all'estinzione anticipata di un contratto di mutuo per l'acquisto della casa; o disapprovare le misure a tutela dei consumatori nei confronti delle assicurazioni per la piena applicazione e l'estensione del *bonus malus*? Altrettanto di difficile comprensione è l'atteggiamento avverso a misure sulla trasparenza nella pubblicità sulle tariffe per il trasporto aereo dei passeggeri e all'informazione degli utenti della rete stradale ed autostradale in relazione ai prezzi del carburante e al traffico sulla rete. Che dire, poi, sulle misure di semplificazione e delle procedure di avvio e di cessazione delle attività imprenditoriali, grazie alle quali ora un imprenditore, un giovane, con una semplice comunicazione inviata, anche per via telematica o su supporto informatico, all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, elimina una serie di adempimenti amministrativi finora previsti, quali l'iscrizione al registro delle imprese, all'INPS, all'INAIL, nonché le pratiche atte all'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. Perché in passato non è stato fatto nulla in merito? Quali sono state le ragioni che hanno impedito di farlo? Infine, quali sono le ragioni che dovrebbero impedire ai giovani di accedere con facilità allo svolgimento di un'attività imprenditoriale e professionale di acconciatore, estetista, pulizia, facchinaggio o guida turistica, per le quali basta ora una semplice dichiarazione di inizio attività da presentare allo sportello unico del Comune competente. Non è accettabile, pertanto, che l'opposizione declami a parole, in tutti i contesti economici e sociali del Paese, il liberismo, la libertà imprenditoriale, la concorrenza e le tutele per tutti i cittadini, quando nei fatti in passato nulla è stato fatto in tal senso e quando, ora, a fronte della sfida lanciata da questo provvedimento non vi è stata una risposta in termini di proposte e di confronto costruttivo. In merito alle misure profondamente criticate dall'opposizione, relative alla scuola, segnalo che le norme introdotte dal provvedimento sono rivolte a fornire maggiori possibilità alla formazione e al futuro dei nostri giovani, con particolare riguardo agli studenti che frequentano gli istituti tecnico-professionali. Ad essi, infatti, viene garantito un sistema di formazione scolastica secondaria adeguato e paragonabile a quello del resto dei paesi comunitari, che consenta loro di completare pienamente la propria formazione e soprattutto di rispondere alle nuove esigenze di preparazione professionale provenienti dal mercato del lavoro. Sulla revoca di alcune concessioni del sistema di Alta Velocità, ricordo che le motivazioni che ci hanno spinto a revocare tali concessioni, che tra l'altro risalgono a circa 15 anni fa, si fondano innanzi tutto sul fatto che le opere oggetto delle concessioni non sono state fatte, ma i loro costi invece sono cresciuti in fase di progettazione sulla base del prezzo iniziale, e che le stesse oggi risultano affidate con procedimenti in contrasto con le regole comunitarie. Pertanto, le accuse che ci vengono formulate, in realtà, sottintendono la volontà dell'opposizione di contrastare il nostro intento di realizzare finalmente tali opere, sulle quali c'è l'accordo di tutta la maggioranza, mediante l'affidamento dei lavori su tratti delle TAV, previsti dal decreto, con il metodo delle gare ad evidenza pubblica, mediante le quali si ristabiliscono i principi di trasparenza e imparzialità ed efficacia economica dell'azione amministrativa, nonché il pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e di quelle contenute nel codice nel codice degli appalti. Sorge il dubbio, pertanto, che forse questo atteggiamento è frutto di una miscela di situazioni irrisolte e irrisolvibili all'interno della Casa delle Libertà; della consapevolezza, innanzi tutto, del fallimento della loro esperienza di governo; delle spinte che da ampi settori del centro-destra muovono alla difesa corporativa di taluni settori imprenditoriali e professionali che vivono di rendita di posizione e lucrano su situazioni anticoncorrenziali a danno di altri, siano essi imprese o cittadini; del tentativo politico, infine, a mio avviso inutile, di impedire la conversione del decreto per argomentare al Paese che non abbiamo un Governo che governa. A questi vostri atteggiamenti confusi e paradossali, colleghi dell'opposizione, noi rispondiamo con la conversione in legge di questo provvedimento, e con questo intendiamo parlare al Paese. Ulteriori motivi che ci spingono ad approvare il provvedimento risiedono nel fatto che esso è parte di una più ampia azione di governo dell'economia nazionale. Il decreto-legge, infatti, si inserisce nel tracciato ambizioso che abbiamo iniziato a disegnare nel luglio scorso, a cui hanno fatto seguito un insieme di altri provvedimenti adottati dal Governo e dalla maggioranza, che nel loro insieme intendono rendere il nostro Paese più dinamico e competitivo. Con il decreto-legge del luglio scorso il Governo ha voluto dare un primo forte segnale al Paese su tale strada e gli interventi lì previsti iniziano ora a produrre i primi apprezzati risultati. Basti pensare a quelli ottenuti con la liberalizzazione della vendita dei medicinali da banco (a seguito della quale i prezzi di quei farmaci si sono ridotti del 20 per cento), con il potenziamento dei servizi dei taxi nelle città, con le nuove regole sui passaggi di proprietà delle autovetture, con l'affermazione e il gradimento che sta ottenendo il risarcimento diretto dei sinistri da parte delle assicurazioni, con l'eliminazione dei costi di chiusura dei conti correnti bancari, con l'apertura di alcune centinaia di nuovi esercizi commerciali. A questo primo provvedimento il Governo ha fatto seguire altre misure per l'allargamento della concorrenza e dei mercati produttivi introdotte nella finanziaria 2007 ed in altri provvedimenti di politica di liberalizzazione dei mercati all'esame del Parlamento e sui quali auspichiamo un'accelerazione nei tempi di approvazione. Ricordo brevemente il disegno di legge delega per il completamento della liberalizzazione dei settori dell'energia, del gas, delle fonti rinnovabili, il disegno di legge per il riordino dei servizi pubblici locali, il disegno di legge per l'introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, delega in materia di professioni intellettuali, il disegno di legge in materia di riassetto delle Autorità indipendenti di regolazione e, infine, il disegno di legge recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali. Nel complesso, questa è una strada che il Governo e la maggioranza hanno imboccato e sulla quale noi gli diciamo di proseguire con grande slancio. Su questo percorso si inserisce a pieno titolo il decreto-legge che stiamo convertendo. Tra l'altro con il lavoro fatto alla Camera sono state accolte modifiche e proposte venute dalle categorie, dalle associazioni interessate e dalla stessa minoranza, a dimostrazione del nostro atteggiamento aperto e concertativo, che però evidentemente non è stato sufficiente a consigliare un atteggiamento diverso da parte del centro-destra, che invece ha messo in moto alla Camera una strategia ostruzionistica, che ha determinato l'allungamento dei tempi di discussione e l'inevitabile necessità di porre il voto di fiducia, al fine di non far scadere il decreto e convertirlo. Cari colleghi, siamo certamente consapevoli che il ricorso al voto di fiducia è uno strumento che riduce in Parlamento gli spazi di dialogo e di confronto fra maggioranza ed opposizione e questo diventa per noi momento serio di riflessione. Ma il rimprovero che ci viene da voi non tiene pienamente conto del fatto che ogni provvedimento, anche quelli che potrebbero dar luogo a confronti costruttivi come questo, in realtà diventano momenti di scontro pregiudiziale. Alla fine di queste considerazioni, annuncio che il Gruppo dell'Ulivo voterà convinto a favore della fiducia, perché, lo ribadisco, il nostro obiettivo è quello di tutelare i cittadini e rendere l'Italia più giusta, più forte e competitiva in Europa e nel mondo.

Abbiamo diverse richieste di voto anticipato, per ragioni anche legate a impegni oggettivi, congressi, eccetera. Utilizziamo questi dieci minuti per anticipare tali richieste dei senatori, cercando di soddisfarle nei limiti del possibile. ***Votazione

avrà luogo mediante votazione nominale con appello. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza. Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. Estraggo a sorte il

Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.